diretta televisiva della RAI. Le prime interrogazioni concernono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'orientamento delle opposizioni circa la partecipazione dell'Italia alla missione in Afghanistan.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Governo italiano ha ribadito l'intenzione di rimanere in Afghanistan e di continuare il proprio impegno, ferma restando la necessità di rivedere la strategia. Contemporaneamente lei, signor Ministro, ha parlato di afganizzazione della nostra azione, nel complesso dell'azione della NATO in Afghanistan. Inoltre, il segretario generale della NATO Rasmussen ha parlato di una nuova visione della strategia, più orientata ad incrementare l'attività civile e

I nostri militari hanno ottenuto in Iraq grandi successi nell'addestramento delle Forze armate e di polizia. Attualmente hanno assunto lo stesso incarico presso le forze afgane. Considerati tutti questi elementi, le chiedo: vi sono ragioni per le quali si dovrebbe mutare la nostra strategia e l'impegno delle nostre forze in ambito afgano? In secondo luogo, sono state adottate disposizioni che integrano

è disponibile a rinforzare la capacità addestrativa dei nostri uomini nei confronti delle forze afgane, anche aumentando il numero degli addestratori che già operano in questa direzione Desidero inoltre esprimere il compiacimento del PdL per la sua iniziativa relativa all'avvio di un'attività che prevede un mese di permanenza di giovani volontari presso le Forze armate, anche perché ciò colma una lacuna

Signor Presidente, signor Ministro, ferma restando naturalmente la libertà che anche al collega Ramponi è riconosciuta di pronunciarsi fuori tema (come si diceva quando eravamo a scuola), mi sembra che stasera siamo qui per parlare - come lei opportunamente ci ha ricordato - delle dichiarazioni rese qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio, nel corso di un *happening* politico-elettorale. fortuna, gli italiani, e non soltanto gli addetti ai lavori, hanno avuto modo, loro malgrado, di avere conoscenza di tali dichiarazioni, intendiamo manifestare tutta la nostra contrarietà ed il nostro disappunto per le affermazioni fatte dal presidente Berlusconi, il quale indiscutibilmente, nel momento in cui ha voluto criminalizzare l'opposizione, ha mentito sapendo di mentire.

determinato un *vulnus* per il nostro contingente, il quale, a causa di quelle dichiarazioni, rischia di sentirsi isolato a livello internazionale e certamente non coperto, come è nella realtà, dal pieno consenso del Parlamento. Allora, signor Ministro, le chiediamo di prendere esplicitamente le distanze dalle affermazioni rese dal Presidente del Consiglio, pregandola anche, senza che questo possa significare coartare la sua volontà, di non dirci che si è spiegato male o che abbiamo capito male.

il Gruppo Italia dei Valori, vera forza di opposizione, ha sempre votato favorevolmente al rifinanziamento delle missioni internazionali, esprimendo criticità sulla modalità sbrigativa con cui veniva liquidata dal Governo una materia tanto importante. La mia parte politica non ha fatto mancare il sostegno ai nostri soldati impegnati all'estero, soprattutto in uno scenario particolare come quello afgano. Vogliamo quindi sapere da lei, signor Ministro, se ritiene che l'opposizione, cioè l'Italia dei Valori, debba vergognarsi per aver chiesto di valutare con attenzione la possibilità di una *exit strategy*. L'Italia dei Valori e i cittadini tutti vogliono sapere da lei, signor Ministro, se ritiene ancora che questa opposizione debba vergognarsi per aver fatto notare che la situazione nel paese afgano è mutata rispetto al 2004 e che, a differenza del passato, oggi siamo in Afghanistan a difesa di un presidente vincitore di elezioni caratterizzate da brogli elettorali.

di assumersi, come Ministro e in qualità di membro del Governo, la responsabilità di garantire la sicurezza dei nostri soldati, quella che ad oggi non avete garantito. Noi dell'Italia dei Valori questa responsabilità ce la siamo assunta con i distinguo e l'attenzione rivolta ai problemi come quelli testé enunciati. Non abbiamo mai bruciato bandiere in piazza e abbiamo sempre votato favorevolmente al rifinanziamento delle missioni, ma abbiamo anche posto il ragionevole dubbio su quale

Signor Presidente, nel corso del comizio di chiusura della Festa nazionale del Popolo della Libertà il Presidente del Consiglio ha attaccato violentemente le opposizioni accusandole di bruciare le bandiere americana ed israeliana e di inneggiare alla morte dei sei soldati italiani in Afghanistan. «A questa opposizione» - ha aggiunto il Capo del Governo - «(...) dico: vergogna, vergogna, vergogna». Le dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi sono false e gravi. Com'è noto, sulle missioni all'estero il Governo ha sempre goduto del sostegno politico e parlamentare delle opposizioni. In particolare, la nostra opposizione moderata, quella dell'Unione di Centro, ha sostenuto senza riserve o condizioni tutte le missioni internazionali, indipendentemente dal colore politico dei Governi che le hanno promosse. Pertanto, in un momento così delicato per il nostro Paese e per i nostri militari impegnati pacificamente in scenari internazionali di guerra, lanciare accuse insensate dividendo artificiosamente l'opinione pubblica è da irresponsabili, così come accreditare l'idea di un Paese diviso sulla politica estera è dannoso per l'interesse nazionale. Da qui l'indignazione dell'UDC e la profonda gratitudine al Capo dello Stato. Il suo intervento è stato veramente provvidenziale per chiarire e recuperare il senso della concordia nazionale. Dopo le parole del Capo lo Stato, però, ci saremmo aspettati un atto forte e formale del Presidente del Consiglio qui in Parlamento, tanto che ne abbiamo fatto espressa richiesta. Siamo quindi qui oggi a conoscere la posizione del Governo, alla luce dei fatti e delle considerazioni espresse in precedenza.

onorevoli senatori per aver posto delle domande che mi danno la possibilità di chiarire e precisare alcune considerazioni. Al di là della rinnovata polemica sulle dichiarazioni del presidente Berlusconi, alla quale comunque non voglio sottrarmi, di anticipare la risposta ai quesiti che mi sembrano più rilevanti. Il quesito più rilevante di tutti mi sembra quello posto, in maniera per la verità strana, dal rappresentante dell'Italia dei Valori, che ha detto testualmente: «Voi non garantite la sicurezza dei nostri militari». Dico al collega di stare tranquillo: la sua preoccupazione - sono contento - è uguale sicuramente alla nostra. Non voglio dire che sia inferiore, ma sicuramente non è superiore alla mia. Posso tranquillizzarla: i mezzi che hanno i nostri militari sono i migliori attualmente esistenti. Il mezzo "Lince" di produzione italiana, che i militari affettuosamente chiamano "San Lince", perché ha salvato

verso la nuova tecnologia non bisogna mai fermarsi, sono attualmente in volo verso l'Afghanistan (e non certo ordinati ora, perché, come sapete, i mezzi militari non si comprano al supermarket, ma in base a una previsione di alcuni mesi fa)

pienamente soddisfatto, a meno che lei non mi dica qual è lo strumento, qual è il mezzo che un soldato, dico anche solo uno, ci ha chiesto e al quale noi non abbiamo cercato di far fronte. Se poi lei pensa che si possa andare a comprare al supermarket ciò che la tecnologia man mano mette in campo, considerando i tempi di produzione, evidentemente siamo su terreni diversi. Il collega Scanu come lei, onorevole Pedica, parlato del problema Berlusconi. Ma voglio prima rispondere all'onorevole Ramponi dicendo che il nostro progetto rimane quello dell'afganizzazione. Siamo convinti, insieme alle organizzazioni internazionali, di dover ritornare. Non è una missione a tempo indeterminato: c'è un momento in cui torneremo, non quando sarà sconfitto il terrorismo, ma quando gli afgani saranno in grado di rispondere autonomamente. Per questo i nostri sforzi, come il senatore Ramponi ha detto, vanno contemporaneamente all'aiuto alle Forze armate ma anche al loro addestramento, perché siano sempre più pronte ed adeguate. Non muta quindi la nostra strategia, non muta l'impiego: man mano che le minacce si fanno diverse, deve aumentare la nostra capacità di risposta e di protezione. ricordo comunque che abbiamo mandato altri due "Predator" ed altri elicotteri "Mangusta", abbiamo autorizzato gli aerei ad una difesa ravvicinata, sia pure senza

di non farvi partecipare i nostri soldati. In quel caso la missione, pur giusta e sacrosanta in termini di principio, cozza infatti contro il nostro desiderio di combattere i talebani e non i *campesinos*, i civili o i contadini che, ahimè, sono quelli che l'oppio lo coltivano. Stiamo cercando con le nostre forze di tentare strade alternative, come quella, ad esempio, di far abbandonare la coltivazione dell'oppio per passare alla coltivazione dello zenzero, obiettivo che nella nostra zona è anche stato

che io e tutto il Governo Berlusconi siamo orgogliosi che il Parlamento, nella sua interezza, abbia dimostrato compattezza nel sostenere i nostri soldati, non soltanto nel momento del dolore ma anche al momento del rifinanziamento delle missioni, pur con le legittime differenziazioni.

a tutti i costi insistere su una polemica che non ha più ragione di esistere, perché è evidente che da parte del presidente Berlusconi, che parlava a braccio, vi è stato un errore nell'uso della terminologia,

è sceso in campo con una dichiarazione apprezzata dallo stesso Berlusconi, da me e da tutto il Governo, insistere su tale polemica (anziché dire che, seppure vi è stato un fraintendimento, siamo tutti uniti nel tutelare i nostri soldati e nel riconoscere che quanto fanno serve a tenere lontano da casa nostra il terrorismo, e non solo ad aiutare l'Afghanistan ma anche a dare più tranquillità alle nostre famiglie) credo sia un errore politico ancor più grave dell'uso, non del tutto appropriato in quella occasione, di quelle parole da parte del presidente Berlusconi.

Userò questi pochi secondi per porre l'accento sull'intenzione di integrare e aumentare le capacità addestrative dei nostri uomini nei confronti dell'Esercito e della Polizia. Questo, dopo i successi che noi abbiamo avuto in Iraq, costituisce un'arma professionale e politica di grandissimo valore in sede internazionale. Sfruttare questa grande occasione che abbiamo è assolutamente commendevole.

che lei ha affrontato, delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ho letto tutte le sue affermazioni non soltanto le sue - che immediatamente hanno voluto ribadire che non c'era alcun intento di colpire l'opposizione. Rimane il fatto però che il presidente del Consiglio, l'onorevole Berlusconi, non abbia ritenuto di dover lui personalmente esprimere il suo pensiero e - se mi consente - le sue scuse nei confronti di un'opposizione che - come lei ha detto - è sempre stata vicino ai soldati che sono impegnati nelle operazioni di supporto alla pace; scuse, soltanto per il fatto che un argomento così delicato, come quello del sostegno ai nostri militari, forse non andava trattato in maniera - se mi consente - propagandistica e non con la leggerezza che in quella circostanza è stata evidenziata. Questa è la mia replica, fermo restando che naturalmente comprendo e

Intanto non ha risposto alla prima domanda, se per lei questa è una missione di pace. Noi siamo tutti uniti per una missione di pace, ma questa non lo è; non lo è, perché lei ha pronunciato, il 28 luglio, queste parole, che in parte risultano anche grottesche: «quello che occorrerebbe, secondo me, sarebbe un aumento a dismisura degli elicotteri». Così ha dichiarato, signor Ministro. Poi ha ammesso: «manca ancora una fase di addestramento specifico e non possiamo rischiare (...) di mandare mezzi per cui i nostri soldati non sono ancora stati addestrati». Questa è la verità, signor Ministro, ed è questo quello che lei in parte ha avuto il coraggio di ammettere. di ammettere. Se il 28 luglio lei ha anche aggiunto che i militari non sono addestrati per usare quei mezzi che dovrebbero garantire la loro sicurezza, e se la sicurezza va garantita perché i talebani ci attaccano in quanto ci avvertono come missione di guerra e non di pace, se la Costituzione ripudia la guerra, se i cittadini italiani non la vogliono..., lascio a lei concludere questo nostro pensiero, signor Ministro. Noi dell'Italia dei Valori lo concludiamo con una sola espressione: *exit strategy*.

e quando si fa riferimento all'opposizione, poiché l'opposizione è solo quella presente in Parlamento nelle sue diverse articolazioni, è in Parlamento che si viene e si chiarisce. Del resto, signor - e concludo - il Capo di un Governo è tale sempre, in pubblico e in privato, e quindi anche durante un comizio, e deve sempre valutare le conseguenze delle sue dichiarazioni, ivi comprese quelle più improvvide e mendaci o, come lei ha confermato oggi, errate. L'Unione di Centro, comunque, continuerà a sostenere le missioni internazionali e i nostri ragazzi, senza se e senza ma,

della Libertà per questa iniziativa, che colma una lacuna lasciata dall'abolizione della leva. Quest'ultima aveva anche una funzione educativa e formativa nei confronti della gioventù maschile italiana,

L'iniziativa del Ministro non fa distinzione: ritiene che possano accedere all'opportunità di passare un mese presso un reparto delle Forze armate come giovani volontari Questo è molto importante. Si tratta di una linea che, devo dire, è già stata seguita, in maniera più o meno analoga, anche dalle Forze armate di altri Paesi che, ad un certo punto, hanno avvertito le conseguenze dall'abolizione del servizio di leva. Signor Ministro, nell'esprimere piena soddisfazione, desidero chiederle se può fare qualche precisazione sull'argomento relativo all'attività di istruzione

dire al collega Ramponi che non intendevo assolutamente interferire nelle sue cose: svolgevo liberamente una mia considerazione, che poi, peraltro, è stata confermata anche dall'intervento del rappresentante della Lega. D'altro canto, come ho cercato di dire poco fa nel mio intervento, verosimilmente le bugie dette dal Presidente del Consiglio erano finalizzate anche a coprire i dissensi che esistevano all'interno sia del Governo che della maggioranza, perché le posizioni della Lega non ce le siamo inventate noi, come non ci siamo inventati neppure i dubbi del ministro Frattini. Ad ogni buon conto, adesso parliamo di precariato. Signor Ministro,

il che significa che già dal primo anno ci sarà una riduzione del personale pari a 4.000-5.000 unità.

la domanda di ingresso nelle Forze armate è infinitamente superiore all'offerta. Offerta che peraltro - ahinoi! - non esiste già promozionale era del tutto assente. Tra l'altro, visto che i soldi non sono bruscolini, la mini naia - 15 giorni per 150 ragazzi - è costata 455.000 euro, con i quali si sarebbero potuti pagare 1.000 soldati veri per 15 giorni. In tempo di vacche morte (neanche vacche magre) 455.000 euro avrebbero svolto un loro ruolo importante!

Lei, signor Ministro, ha dichiarato con orgoglio che la mini naja può rappresentare, per i giovani che vi hanno partecipato, l'occasione di verificare sul campo che cosa è la vita militare, ma ha pure affermato che tra gli intenti di tale iniziativa ci sarebbe anche quello di colmare il vuoto che si è creato da quando si è passati ad un modello di esercito composto esclusivamente di professionisti. Sappiamo bene che la crisi del reclutamento nelle Forze armate è dipesa dai tagli al bilancio della Difesa e non da una diminuzione delle domande di arruolamento, che, anzi, sono maggiori di quanto le Forze armate stesse possano permettersi di soddisfare. La domanda che le pongo dunque, è questa: non sarà stata, quella della mini naja, un'altra iniziativa propagandistica? Se i tagli del bilancio hanno aggravato anche le ordinarie attività del personale della Difesa, è lecito pensare che non si è in grado di garantire un concreto inserimento ai giovani che hanno voluto partecipare alla mini naja, e quindi che si sia pensato di coinvolgerli solo a scopo pubblicitario, il che, tenuto conto della condizione dei tanti, troppi precari delle Forze amate, apparirebbe del tutto irrispettoso nei loro confronti.

ha affrontato, in alcune mozioni presentate dai colleghi dei Gruppi parlamentari dell'opposizione, il tema della difesa, del processo di attuazione del Nuovo modello di difesa e della difficoltà, rappresentata dai vertici militari in diverse audizioni tenute in Senato,

(ce li hanno appena consegnati). Non mandiamo nuovi mezzi a soldati che non li hanno prima testati in Italia: prima di mandarli bisogna che si addestrino in Italia; non li facciamo provare in mezzo al pericolo. Questo mi sembrava

al servizio militare a tempo prefissato o a tempo indeterminato. Al contrario, la *ratio* della mini naja è esattamente opposta:

professionalmente il militare, ma vogliono avere una vicinanza con i valori che promanano dalle Forze armate, primo tra tutti l'amore per la Patria, ma anche

che prima avevano la linfa dei giovani di leva, e che oggi non hanno più. Abbiamo iniziato con gli alpini, che non hanno più quell'afflusso di giovani, provenienti soprattutto dalle valli,

mentre non c'è nessun problema per gli ufficiali dei Carabinieri che ieri hanno protestato qui davanti, perché tutti saranno inseriti (spero lo stesso avvenga anche per gli ufficiali della Marina che pure erano a manifestare), per i militari in ferma breve la questione esiste

un equilibrio tra le spese per l'investimento e quelle per l'addestramento e per il reclutamento. Ieri mi è stato portato alla firma un un accordo con la Francia che prevede una risorsa aggiuntiva per la costruzione da un minimo di sei a un massimo di dieci fregate italiane, oltre a quelle francesi. Prima di

ma l'idea portante è che è inutile ridurre al massimo il numero dei militari se poi ci impegniamo (non voglio dire che sia così per le fregate, ma in assoluto) per la che eccedono la possibilità di utilizzo. Se non abbiamo poi le risorse per tenerle in addestramento, allora vediamo di privilegiare - questa è la mia linea, ve lo assicuro - prima di tutto l'elemento umano delle Forze armate. armate. Le nostre Forze armate devono essere dotate delle migliori attrezzature, devono avere le migliori navi e i migliori aerei, ma se non avessero i migliori militari, con le forti motivazioni morali che hanno oggi, che tanti risultati anche d'orgoglio ci danno, oltre che di sacrificio, sarebbero assolutamente lontane lontane da quello che noi desideriamo. Questo è il mio impegno e sarò pronto, come sempre, nelle sedi competenti (come le Commissioni riunite) a dare dettagli e informazioni specifiche, come ho sempre fatto, circa la possibilità di ridurre al minimo o addirittura di azzerare

Il problema cruciale resta grave e irrisolto. Tantissimi giovani sono già entrati nelle Forze armate come volontari, dedicando loro anni della loro vita, con l'obiettivo di formarsi al meglio e con il sogno di essere stabilizzati. Eppure, a causa dei tagli apportati dal suo Governo al bilancio della Difesa, a questi giovani ancora non è data la possibilità di divenire stabilmente membri delle nostre Forze armate. Le vorrei ricordare, appunto, le migliaia di volontari in ferma prefissata - così come lei li ha definiti, signor Ministro - che ogni anno cercano una stabilizzazione e le centinaia di giovani laureati che frequentano i corsi di allievi ufficiali in ferma prefissata e che, dopo quattro anni dedicati alla Nazione, si ritrovano in mezzo a una strada. non faccia credere che la mini naja sia volta semplicemente ad avvicinare i giovani alle Forze armate. In realtà, ha comportato uno spreco di risorse e una distrazione delle stesse professionalità, che sarebbe stato più coscienzioso destinare altrimenti.

è funzionale all'avvicinamento dei giovani al mondo delle Forze armate, alla conoscenza delle istituzioni, al rispetto e alla condivisione dei valori della nostra Costituzione democratica e repubblicana, all'amore per la Patria. Quanto alla vicenda dei tagli al bilancio della Difesa, le faremo avere i resoconti parlamentari sulle denunce dei vertici militari in ordine a tali ristrettezze. Per la verità, con molta onestà, capisco dalle sue parole che il reclutamento è in crisi e che anche per la Difesa, come per la scuola e l'università, il futuro del Nuovo modello di difesa è affidato più al Ministro dell'economia che al Parlamento che al Parlamento e al Ministro della difesa. Evitiamo però che la naja breve diventi l'ennesima foglia di fico dietro cui nascondere le carenze economiche e strutturali della Difesa, così come le ronde e i militari per le strade sono la foglia di fico per nascondere le carenze di organico di Polizia e Carabinieri.

Onorevoli colleghi, come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, l'esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze avrà luogo martedì 6 ottobre, alle 16, anziché alle ore 12. Pertanto, la seduta antimeridiana non avrà luogo.